Colleghi, è di ieri la dolorosa notizia della morte del tenente Massimo Ranzani e del ferimento di altri quattro alpini appartenenti al 5° Reggimento Alpini, impegnato in missione in Afghanistan. Non appena appresa la notizia, il presidente Schifani ha rinnovato i sentimenti del più profondo e affettuoso cordoglio, suo personale

sempre più spesso sottoposti ad attacchi nelle missioni internazionali di pace in cui sono impegnati. Il loro lavoro è fondamentale per l'affermazione della democrazia e l'aiuto alle popolazioni civili dei Paesi ove sono dislocati, in particolare dell'Afghanistan. Il ministro della difesa, onorevole La Russa, riferirà domani in Aula, alle ore 16,30, su questo tragico episodio. In segno di lutto e di vicinanza ai familiari dei soldati colpiti, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

Antonio Landolfi era un socialista riformista, fu stretto collaboratore di Giacomo Mancini, sia quando Mancini era Ministro e guidava il Partito socialista italiano sia quando entrò nella sua fase calante. Landolfi capì, senza reticenze ideologiche, la novità politica dell'avvento di Bettino Craxi; accompagnò il percorso di Craxi senza mai intrupparsi tra gli apologeti del capo: mai cortigiano, mai adulatore. Egli lottò sempre per un socialismo liberale, in un Paese che socialdemocratico e liberale non era, ma che aveva largamente preferito le chiese ideologiche e le scorciatoie del consociativismo. Scrisse molto di storia della cultura socialista, di garantismo, ed ebbe modo di intervenire spesso su importanti riviste, come «Mondo operaio» e «Le ragioni del socialismo». Così ha vissuto, sino alla fine dei suoi giorni. A lui va il ricordo affettuoso, spero, di tutto il Senato; alla moglie, alle figlie e alla nipotina un abbraccio fraterno

al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 10 marzo prossimo. Fermi restando gli argomenti già previsti, il calendario della settimana corrente potrà essere integrato con la deliberazione dell'Assemblea sulla costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione promosso dalla corte d'appello di Roma. La seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 10 in relazione alla convocazione delle Commissioni congiunte 1a e 3a di Camera e Senato, presso la sede della Camera dei deputati, per un'audizione del Ministro dell'interno sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi del Nord Africa. Domani, alle ore 16,30, come ho già detto, il Ministro della difesa renderà un'informativa sulla morte di un militare del contingente italiano in Afghanistan e sul ferimento di altri militari. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno. Nel pomeriggio di martedì 8 marzo sarà discusso il disegno di legge sulle modifiche al codice di procedura penale a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, già approvato dalla Camera dei deputati. La seduta pomeridiana di martedì 8 marzo avrà inizio alle ore 18, a conclusione della cerimonia di inaugurazione della nuova sala Koch in occasione della Festa della donna. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre l'esame di mozioni sulla situazione dei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, anche con riferimento ai flussi migratori, mozioni della senatrice Franco Vittoria ed altre connesse su donne e sistema dei *media*, nonché del disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione, ove concluso dalla Commissione. Infine, la Conferenza dei Capigruppo la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della lettera con la quale, in data odierna, il senatore Viespoli ha preannunciato l'imminente costituzione di un nuovo Gruppo parlamentare, composto da dieci senatori, comprendente tre senatori provenienti dal Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia. Pertanto, la Conferenza dei Capigruppo ha altresì preso atto che, non appena formalizzati i predetti adempimenti, il Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia dovrà considerarsi sciolto, ai sensi dell'articolo 14, comma 16, del Regolamento.

nonché dell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi

di negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria con il documento in titolo in ordine alle intercettazioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4 dell'informativa CC-RONO-RC del 10 dicembre 2007; *b)* di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

casuali non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva (nel qual caso si rientra nella fattispecie dell'articolo 4

in questione, configurata come uno strumento di controllo parlamentare sulle eventuali violazioni surrettizie della norma costituzionale.

dei carabinieri di Reggio Calabria datata 10 dicembre 2007) si afferma, anche da parte del relatore e dell'attuale maggioranza, il carattere casuale dell'intercettazione in questione, nonchè di quelle relative ai due fax.

che soprattutto con le valutazioni e le indicazioni della Corte costituzionale, perché si opererebbe una sorta di invasione di campo nell'autonomia di valutazione dell'autorità giudiziaria.

tre casi venga concessa l'autorizzazione alla magistratura per utilizzare questi atti. Negli altri casi, trattandosi di intercettazioni non casuali,

in senso contrario alla proposta della Giunta per un discorso di politica generale in materia di attività investigative. Noi non finiremo mai di denunziare l'ipocrisia della legge n. 140 del 2003. In virtù di tale legge, non si vietano le intercettazioni nei confronti dei parlamentari, ma si dice che esse sono legittime e possono essere fatte soltanto dopo aver chiesto l'autorizzazione alla Camera di appartenenza. Ora, è all'evidenza una clamorosa ipocrisia: è come dire che le intercettazioni nei confronti dei parlamentari non debbano farsi, perché prima di poterle fare bisogna svolgere un'istruttoria e un dibattito che può durare anche mesi (nel nostro caso andiamo avanti da sette-otto mesi); si fa un dibattito e, ove ne esistano i presupposti, si dice al collega parlamentare che si autorizzano le intercettazioni della sua utenza. È un'ipocrisia. Noi denunziamo questa ipocrisia votando contro la proposta della Giunta che è ancorata alla *ratio* profonda,

Signor Presidente, egregi colleghi, non credo che sull'argomento abbiamo necessità di sviluppare un ragionamento ad ulteriore sostegno di quanto già sostenuto dal relatore e approvato nella Giunta delle elezioni

nel fatto in sé e per sé che emerge dal tenore delle conversazioni intercettate, e che è la non configurabilità di qualsiasi ipotesi di abuso della potestà funzionale, indispensabile per affermare la ricorrenza del *metus publicae potestatis*. Soprattutto, mi soffermerei sul fatto che la Giunta ha proposto di confermare quanto già aveva formulato nella seduta del 7 ottobre 2009 anche alla luce del del ragionamento che aveva seguito la Corte costituzionale con le sentenze nn. 113 e 114 del 2010, è stato assolutamente confermato l'assunto già approvato dalla Giunta. del 2007. L'intercettazione del parlamentare - dicevo prima - per essere casuale deve essere imprevista, e solamente in questo caso si può sanare attraverso l'autorizzazione del Parlamento fornita pertanto, che, seppur approvata soltanto a maggioranza all'interno della Giunta, quest'Aula parlamentare possa senz'altro confermare la proposta del relatore Sarro e negare l'autorizzazione richiesta dall'autorità giudiziaria. Grazie,

già deliberato dalla Giunta con riferimento specificatamente alle intercettazioni delle comunicazioni dell'ex senatore Fuda. Esse ribadiscono, infatti, la definizione di casualità già fissata dalla sentenza n. 390 del 2007. L'intercettazione del parlamentare - dicevo prima - per essere casuale deve essere imprevista, e solamente in questo caso si può sanare attraverso l'autorizzazione del Parlamento fornita *ex post*. ha ragione, Presidente, quando ci richiama a cercare di avere un tono di voce tale da consentire almeno di ascoltare noi stessi quando parliamo.

della norma che prevede la richiesta di autorizzazione per l'utilizzazione delle intercettazioni con riferimento alla sua applicazione nei confronti del parlamentare (diversamente appunto da quanto ha stabilito per la fattispecie in cui le intercettazioni contengano elementi di prova contro terzi). Pertanto, sulla base di queste considerazioni,

Grazie, di restituire gli atti all'autorità giudiziaria per le restanti intercettazioni, nel presupposto che queste ultime non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ma direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Come Partito Democratico, di fronte ad una vicenda come questa, che riguarda un'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche e di fax, riteniamo di dover utilizzare il nostro senso di responsabilità, senza assumere posizioni ideologiche o ideologizzate.

Qui ci troviamo di fronte ad intercettazioni sicuramente casuali; questo è stato detto e sostenuto anche dall'attuale maggioranza in sede di Giunta, tanto che è stato scritto che la maggior parte delle intercettazioni oggetto del documento hanno avuto carattere casuale. In questo caso, la legge e la Corte costituzionale dicono che dovrebbero essere pacifici il nostro nulla osta il nostro consenso autorizzativo nei confronti della richiesta dell'autorità giudiziaria. Invece, per le intercettazioni che non sono casuali, è corretta l'indicazione di rigetto della richiesta dell'autorità giudiziaria.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ritenendo che non ricorrano i presupposti per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Grillo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Chiedo al relatore, senatore Balboni, se intende intervenire.

Gli argomenti sono elencati nella relazione scritta depositata agli atti: mi permetto soltanto di ricordare che queste intercettazioni, iniziate casualmente, in modo indiretto, su altre utenze, si sono poi concretizzate su utenze del Senato della Repubblica. Credo non vi sia dubbio alcuno

la richiesta di autorizzazione alla sua utilizzazione, mi sembra un argomento quantomeno singolare. Una minima diligenza avrebbe dovuto indurre gli inquirenti ad approfondire a chi effettivamente corrispondesse quella determinata utenza del Senato della Repubblica e, se lo avessero fatto - come secondo me era loro dovere - avrebbero scoperto che corrispondeva ad un senatore, il quale tra l'altro, nello stesso periodo, aveva assunto posizioni pubbliche inequivocabili proprio sugli argomenti sui quali in quel momento stava indagando l'autorità giudiziaria. Mi permetto di ricordare all'Assemblea che, nei giorni scorsi, lo stesso procuratore della Repubblica che ha chiesto l'autorizzazione a utilizzare le intercettazioni ha rassegnato le sue conclusioni nel corso del procedimento penale

Il senatore Balboni propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, in quanto le intercettazioni avrebbero dovuto essere sottoposte alla procedura di cui all'articolo 4 della

del Senato, scorporandolo dal nesso funzionale, che evidentemente esula dall'ambito pertinenziale connesso alla funzione e quindi rischia di portarci su un terreno in cui la guarentigia verrebbe interpretata in modo tale da rendere impraticabile l'utilizzo della medesima.

Grazie, dell'atto di indagine». Se tale atto è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. dunque, la lettera della sentenza della Corte costituzionale, che tutti citiamo perché è quella che ha aiutato ad interpretare tale disposizione.

la lettera della sentenza è inequivocabile. Quindi, nel caso che stiamo esaminando, come negli altri che si sono presentati o che si potranno presentare, il criterio cui ci dobbiamo attenere in ordine agli atti di cui stiamo parlando è particolarmente stringente, in quanto non possiamo fermarci al fatto che, in astratto, fosse prevedibile che l'intercettato si relazionasse con il parlamentare: occorre che, in concreto, il magistrato richiedente l'intercettazione avesse previsto che l'intercettato si sarebbe relazionato con il parlamentare. In caso contrario, abbiamo delle intercettazioni meramente fortuite, e ci comportiamo quindi come ha ricordato prima il collega Casson. Noi dobbiamo valutare una richiesta di utilizzazione di 35 intercettazioni telefoniche che si sono svolte dal 26 giugno al 28 luglio 2005. Il relatore le ritiene tutte svolte illegittimamente, in quanto prive di una preventiva autorizzazione, mentre il giudice richiedente le ritiene tutte svolte legittimamente e non necessitanti di una precedente precedente autorizzazione, in quanto tutte fortuite. Questo è il punto su cui credo ci si debba soffermare, sia perché questo caso è particolarmente significativo,

Richiamo a questo riguardo un'ulteriore sentenza, molto recente, della Corte costituzionale, proprio perché tali intercettazioni si svolgono in un arco temporale vasto. Mi riferisco alla sentenza costituzionale del 2010 sul caso Pecoraro Scanio, che è significativa, perché prende in considerazione, trattando dell'occasionalità delle intercettazioni, il caso in cui le intercettazioni siano articolate nel tempo, e quindi la verifica della loro occasionalità - ci ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 113 dello scorso anno - «deve farsi, di necessità, particolarmente stringente». Ricordo a tutti che la sentenza dice che ove «nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: nel senso che (...) le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali.

Ci sono stati restituiti gli atti: il giudice si è limitato a dirci che il senatore Grillo non era né formalmente né sostanzialmente indagato nel procedimento che diede luogo a delle intercettazioni;

fatti che abbiamo riscontrato. Nella sequenza delle 35 intercettazioni telefoniche risulta chiaramente che, a decorrere dal 14 luglio 2005, in una conversazione intercettata tra

Grazie,

ricadono sotto l'ambito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione le conversazioni intercettate dalla ventiseiesima alla trentacinquesima, quindi a far seguito dalla data che abbiamo ricordato in cui c'è evidenza in atti del titolare dell'utenza, in quanto

Grazie,

e che, se riferita all'intestazione dell'utenza telefonica, rischia di estendere la guarentigia persino a soggetti non tutelati dall'articolo 68 della Costituzione.

che quel numero riguardava un senatore in carica, richiedendo che il dato emergesse dalla relativa anagrafica. Se così fosse stato, nessuno avrebbe intercettato il senatore Grillo.

la tesi che ora si sostiene è che il senatore Grillo non era persona indagata, ma poiché vennero intercettate delle telefonate su un'utenza intestata al Senato della Repubblica, era consequenziale il fatto che che l'utente dovesse essere un senatore della Repubblica. Francamente questa mi sembra un'affermazione destituita di fondamento,

una volta scoperto il fatto che l'utenza era del Senato della Repubblica, avrebbe dovuto

il convincimento del magistrato è stato così forte da non tener conto del rispetto della legge, oppure siamo di fronte ad un convincimento aprioristico rispetto al problema?

Il fatto che l'utenza fosse indirettamente intestata al Senato avrebbe dovuto indurre l'autorità giudiziaria, proprio perché vi poteva essere il dubbio della provenienza dell'utilizzatore del telefono, ad accertare il fatto,

o l'intestazione del telefono di provenienza e si commettono errori. Questa è superficialità, ma l'obiettivo era di intercettare senza essere autorizzati. Ecco allora il motivo per cui abbiamo la ferma volontà determinata convinzione di votare per la conferma della decisione adottata dalla Giunta delle elezioni

nel 2005 mancanza di rispetto della norma da parte dei magistrati. Noi ora stiamo leggendo le vicende del 2005 con gli occhiali del 2010-2011,

stabilizzati. Quindi, quella vicenda si era sviluppata in una fase in cui le coordinate applicative offerte dalla normativa erano dubbie, tant'è vero che poi vi è stata una declaratoria di illegittimità costituzionale da parte della

che, come relatore, non accetto la proposta formulata dalla senatrice Leddi, non perché io non sia d'accordo con lei, ma perché proceduralmente la Presidenza ci informa che non è possibile.

era intestata al Senato nel senso che veniva addebitato l'utilizzo al Senato, ma era il cellulare del senatore Grillo. Stiamo parlando, cioè, di un'intercettazione sull'utenza telefonica del cellulare del senatore Grillo, che risulta intestato al Senato perché Grillo lo utilizzava

d'accordo Presidente, alla luce del dibattito che c'è stato, per le motivazioni tecniche dette, il Gruppo del Partito Democratico si asterrà in questa votazione, ribadendo comunque che, alla luce della nostra analisi, alcune intercettazioni erano assolutamente illegittime; altre, per le ragioni dette, no, a prescindere dall'utenza.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del signor Giovanni concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Chiedo al relatore, senatore Sarro, se intende intervenire. *relatore*. Signora Presidente, rimettendomi alla relazione per la ricostruzione della vicenda sulla quale la Giunta si è pronunciata e anche per quanto riguarda le conclusioni che sono state rassegnate, mi preme in questo caso rimarcare come quanto accaduto all'allora senatore Giovanni Battaglia, a proposito di quella che è un'attività tipica del parlamentare, cioè l'esercizio del diritto di critica e dell'attività di denuncia rispetto ad una situazione estremamente pesante, come quella che ha originato questa vicenda - vale a dire la denuncia sul mancato accertamento della responsabilità in ordine all'omicidio del giornalista Spampinato, quindi anche una critica molto forte espressa dal senatore

di atti tipici, che pure ricorrono nel caso di specie: precedentemente vi era stata da parte dello stesso parlamentare, nell'esercizio della funzione di sindacato ispettivo,

nell'esprimere le proprie opinioni, rendersi interprete anche di un disagio e di una difficoltà che un'intera comunità, come quella di Ragusa nel caso di specie, aveva in più occasioni soprattutto occasioni pubbliche, commemorative - manifestato per il mancato accertamento delle responsabilità e dell'identità degli esecutori di un omicidio così importante.

è proprio del parlamentare l'esercizio del diritto di critica e di denuncia, azioni che possono essere sicuramente qualificate come tipiche della funzione parlamentare. Ribadisco naturalmente che le conclusioni in ordine all'affermazione dell'insindacabilità,

ha comunicato che, nella seduta del 1° marzo 2011, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le dichiara valide: per la Regione Umbria, Francesco Ferrante; per la Regione Campania, Franco Cardiello; per la Regione Sicilia, Maria Giuseppa Castiglione. Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni onorevoli colleghi,

senatore D'Ambrosio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Signora Presidente, credo che la mancanza d'interesse sia dovuta anche al fatto che questo disegno di legge fu già approvato nella passata legislatura qui in Senato pressoché all'unanimità.

è stata imposta dalla necessità di combattere meglio la criminalità organizzata e, in particolare, la criminalità transfrontaliera.

forza alla lotta alla criminalità transnazionale e, soprattutto, alla lotta alla criminalità organizzata attraverso l'istituzione di squadre

il secondo, addirittura il testo di legge che fu poi approvato in Senato.

che fu approvato nella scorsa legislatura, perché, mentre nella scorsa legislatura si pensò di inserire le norme relative all'istituzione delle squadre

questa lotta a distanza e per attuare anche in Italia le squadre comuni investigative,

Nell'articolo 2 si disciplina la costituzione di queste squadre da parte del procuratore della Repubblica, direttamente o su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera, quando vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse nel territorio di più Stati o di assicurare il loro coordinamento e queste indagini siano relative ai delitti

quando si tratta di indagini particolarmente complesse, anche se non sono relative a delitti di questa gravità, purché siano punite con pena massima non inferiore ai quattro anni, ugualmente possano essere costituite le squadre comuni sovranazionali. Naturalmente, si è previsto anche che, allorché la richiesta di costituzione provenga da un'autorità straniera, il procuratore competente la trasmetta immediatamente, senza ritardo, al Ministro della giustizia, il quale entro dieci giorni può disporre che ad essa non sia dato corso qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi

la costituzione della squadra e la nomina dell'ufficiale di polizia giudiziaria che la dirige, nonché la sua durata. L'articolo 4 riguarda i poteri e la facoltà dei membri distaccati dei rappresentanti e degli esperti stranieri. La direzione delle indagini resta - così com'è previsto dal codice di procedura penale - al pubblico ministero e viene anche stabilita la possibilità di vietare, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, l'utilizzazione delle informazioni investigative da parte dell'autorità straniera quando si potrebbero compromettere le indagini. L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni provocati dai componenti stranieri Grazie nell'adempimento dei compiti delle squadre comuni sovranazionali risponda sempre lo Stato, salva la possibilità poi di fare una rivalsa nei confronti dello Stato cui appartiene il membro della squadra.

strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, senza alcun ulteriore onere per lo Stato. Naturalmente il fatto stesso che il il testo che viene sottoposto oggi all'esame e all'approvazione dell'Assemblea sia il risultato del lavoro di un Comitato ristretto nell'ambito della Commissione e sia stato approvato all'unanimità ha comportato che siano stati presentati pochissimi emendamenti, alcuni dei quali inviterei a ritirare (mi riferisco a quelli del senatore Li Gotti), mentre per altri

tutto sommato gli stessi. Si giunge a un importante risultato con uno strumento di grande interesse nella lotta al crimine, che aiuta moltissimo a superare le difficoltà che spesso si creano in materia di rogatorie per il compimento di singoli atti.

dal rischio di offesa criminale indubbiamente facilita le indagini, in un coordinamento disciplinato dalle norme codicistiche e, quindi, è un aiuto concreto nella lotta al crimine.

ora mancheranno alcuni altri provvedimenti che seguimmo, quando si lavorava al Ministero della giustizia, nella fase

di dover collocare all'esterno del codice di procedura penale degli strumenti investigativi che sono disciplinati dal codice di procedura penale e che ad esso si riferiscono. Poiché il nostro codice di procedura penale disciplina le rogatorie attive e passive, cioè quando noi le richiediamo

indagini fatte congiuntamente ad altre polizie, ma su fattispecie di reato di interesse del nostro Paese,

modificando o integrando il codice con nuovi istituti. Non ne capisco la ragione; ad ogni modo, nella sostanza non cambia nulla. Gli emendamenti che il nostro Gruppo aveva presentato erano indirizzati soltanto a ribadire questa collocazione

Peraltro, i Paesi membri dell'Unione europea rivolgono spesso all'Italia accuse di scarsa attenzione agli Accordi internazionali ed in effetti è grave il ritardo con cui il Parlamento ratifica Convenzioni ed Accordi internazionali. Moltissime sono le convenzioni in attesa di ratifica. Secondo il procuratore nazionale antimafia, «questa mancanza spesso intralcia la collaborazione con altri Paesi, che invece a ciò hanno provveduto e limita la creazione di nuove strutture operative (esempio le squadre investigative comuni), che in Europa sono state pensate per superare i vecchi formalismi delle tradizionali rogatorie internazionali». In effetti, in merito alla cooperazione internazionale, la Commissione antimafia ha dovuto registrare il grido di allarme del rappresentante nazionale per l'Italia che fa funzioni presso Eurojust, la dottoressa Manfredda, nell'audizione del 22 aprile 2009, ha voluto ricordare che «l'Italia purtroppo è in forte ritardo nelle attività di implementazione di gran parte delle decisioni e delle decisioni quadro fondate sul principio del mutuo riconoscimento» e che «l'attuazione delle decisioni sta diventando sempre più un momento fondamentale, una sorta di cartina di tornasole che fa emergere i possibili conflitti di giurisdizione e che consente anche di prevenirli». alla luce di questi elementi, noi salutiamo con particolare attenzione e soddisfazione il fatto che le squadre investigative comuni possano finalmente diventare una realtà. La squadra investigativa comune rappresenta infatti una nuova figura di cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri dell'Unione europea, che può coinvolgere non solo autorità giudiziarie e di polizia, ma anche quelle autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode

ma piuttosto individuare uno specifico ambito di azione comune che consenta di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale. Un intervento normativo interno è necessario per dare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alle disposizioni sulle squadre investigative comuni: e come già hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, durante la XV legislatura il Senato della Repubblica aveva approvato con modifiche l'Atto Senato n.

Il provvedimento dell'epoca conteneva alcune novelle al codice di procedura penale, che il senatore Li Gotti ha in precedenza richiamato; il provvedimento attuale ha una diversa collocazione rispetto al codice di procedura penale, ma in buona sostanza riproduce il disegno di legge del precedente Governo e quanto già approvato dall'Assemblea del Senato nella precedente legislatura. legislatura. La Commissione parlamentare antimafia ha spesso posto l'attenzione sulla necessità di procedere con celerità all'attuazione della normativa sulle squadre investigative comuni:

atto. L'auspicio che si potesse procedere finalmente a una calendarizzazione in Assemblea del provvedimento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato ha però trovato accoglimento e quindi noi, con grande soddisfazione - trattandosi di un disegno di legge presentato dal precedente Governo,

pur avendo una normativa d'eccezione per quanto riguarda il contrasto al crimine organizzato e al terrorismo. *(Applausi del

Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, anch'io segnalo che questo disegno di legge arriva tardi e ogni ritardo nella lotta alle mafie causa dei danni, spesso irreparabili.

scelto l'Italia per realizzare la prima convenzione internazionale sulla lotta alle mafie - mi riferisco all'incontro tenutosi alla fine del 2000, ovvero 11 anni fa fa - proprio perché il nostro Paese ha una cultura giuridica, un insieme di norme e di strumenti nella lotta alle mafie, che sono il prodotto della fatica e della morte di tanti servitori dello Stato, ha raffinato, grazie a questa dolorosissima esperienza, una serie di strategie antimafia da segnalare alla comunità internazionale.

per le indagini internazionali contro le mafie e - non dimentichiamolo mai - il terrorismo. Come voi sapete, l'impellenza che sottolineava l'ONU è dovuta al fatto che le organizzazioni mafiose più il modello italiano: pensate un po' alla 'ndrangheta che, oltre a cosa nostra e alla camorra, è diventata una delle organizzazioni più importanti al mondo. La specificità delle mafie italiane è che sono molto territoriali, sono in grado addirittura di intervenire su un microcosmo come quello di quartiere, e nello stesso tempo sono iperglobalizzate, potendo intervenire su scala internazionale in tempo reale.

ed è capace di mettere a disposizione di tali cartelli il servizio del riciclaggio, con professionalità che ha costruito al proprio interno. Ecco perché l'ONU ha individuato la necessità delle squadre comuni per le indagini internazionali. Il paradosso sta nel fatto che l'ONU trae dall'Italia tale indicazione e suggerisce agli altri Paesi di normare in questo campo; i trattati vengono poi sottoscritti da molti Paesi, che li recepiscono, senza avere la cultura giuridica antimafia, con delle innovazioni senza precedenti all'interno dei loro ordinamenti, mentre l'Italia non lo fa,

che svela anche l'ipocrisia di un Governo che sbandiera, un giorno sì e un giorno no, i grandi successi del nostro Paese nella lotta alle mafie.

Anche a me fa specie che abbiamo utilizzato una legge speciale. Ricordo a tutti, e al Governo, che ancora manca un grande appuntamento, anzi due: uno concerne una legge che non è stata ancora realizzata, quella sull'autoriciclaggio,

contestualmente di volerla portare a termine. Eppure troviamo ancora ostilità da parte di chi dovrebbe essere soddisfatto nel vedere che esiste ancora un po' di cooperazione in quest'Aula, e non solo contrapposizione. È vero che il periodo è stato lungo: questo atto arriva dopo lavori che partono da lontano, da un percorso che parte probabilmente dal 1999, poiché

Stati membri si adeguino alle disposizioni, fissando la necessità di combattere tutte le forme di reati connessi alla criminalità organizzata. Noi siamo stati estremamente corretti e onesti, e abbiamo riconosciuto che il Governo Prodi si era già attivato in questo senso. Infatti, solo la legislatura che si è chiusa anticipatamente non ha permesso di portare a termine l'Atto

collaborazioni ai fini della repressione dei reati più gravi, che sono quelli collegati alla criminalità organizzata. Per la prima volta, inoltre, si parla di sicurezza internazionale: si percepisce che ogni Stato da solo argina appena quanto succede in casa propria, ma esiste un sistema di criminalità che va affrontato in un contesto di collaborazione e cooperazione internazionale. Ci siamo già dotati, come richiedeva il Trattato di Prüm, della banca dati dei DNA, che è importantissima perché consentirà con estrema velocità e certezza l'identificazione delle persone che commetteranno reati.

Non ce ne accorgiamo (e questo è un bene), ma adesso voliamo più sicuri, perché sono state introdotte delle scorte armate su ogni volo di linea.

(pensiamo alle grandi organizzazioni transnazionali che operano nel settore del traffico degli stupefacenti). Se cambia la criminalità, non c'è dubbio che gli Stati debbano reagire di conseguenza e trovare forme di cooperazione maggiore tra organismi,

sollevato prima, il grosso dei problemi con cui avremo sempre più a che fare sarà il terrorismo internazionale. Già qualcosa è stato fatto: non possiamo dimenticare l'Ufficio europeo

una nuova figura e probabilmente diventeranno anche la punta di diamante della cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo.

in termini di politica estera, si trovi un minimo comun denominatore, un ragionamento che abbia come base gli interessi del nostro Paese.

nostro cittadino, di qualsiasi colorazione politica esso sia. I cittadini hanno soltanto bisogno di maggiore sicurezza, e queste Aule, e noi nel nostro piccolo, abbiamo solo l'obbligo di dare questo tipo di risposta.

Signora Presidente, nel giorno del funerale ritengo doveroso ricordare in quest'Aula l'onorevole Alcide Berloffa, scomparso l'altro ieri a Bolzano all'età di 88 anni. Nato a Trento nel 1922, fu giovanissimo consigliere comunale a Bolzano (dove la famiglia si era trasferita) e deputato ininterrottamente dal 1953 al 1968 e, poi, dal 1972 al 1976. Ricordare Alcide Berloffa significa ripercorrere il lungo cammino compiuto dall'Alto Adige/Südtirol dopo la seconda guerra mondiale, fino alle attuali avanzate forme di speciale autonomia che garantiscono a quella Provincia, nel quadro della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il mantenimento di un buon grado di convivenza ed integrazione fra i diversi gruppi linguistici. Infatti, Alcide Berloffa fu interlocutore appassionato, rigoroso e lungimirante sia della classe politica dirigente locale (con il presidente Silvius Magnago mantenne un peculiare rapporto), sia della classe politica dirigente nazionale (dal presidente De Gasperi al presidente Moro, al presidente Andreotti). Determinante fu il suo apporto alla predisposizione del cosiddetto Pacchetto che sfociò nel nuovo statuto di autonomia del 1972 e, infine, nella «quietanza liberatoria»

impostando ed approvando diecine di norme di attuazione, che contribuirono a configurare compiutamente l'autonomia speciale di quelle terre di confine. Come tutti i costruttori istituzionali, fu forse più rispettato che amato, ma nel momento sintetico della morte non possiamo che apprezzare profondamente il suo impegno politico di risolutore di conflitti e di pertinace ricercatore di vie istituzionalmente più corrette ed aggiornate per la valorizzazione delle diversità nel quadro nazionale.

riguarda il fenomeno dell'occupazione ovvero autogestione delle scuole, un fenomeno che potrà avere anche dei risvolti positivi - che però a me sfuggono ma che fa perdere settimane di lezione a molti allievi, mettendoli nelle condizioni di non poter usufruire del diritto all'istruzione garantito dalla Costituzione,

alzare ulteriormente il volume, oltre ad essere contraria a norme solennemente approvate anche in quest'Aula, non risolve il problema, perché anche chi ha bisogno di conferire, sia pure brevemente (e a volte anche non brevemente) con il vicino, il Capogruppo o un collega